L'inizio delle vicende relative alle aziende citate negli atti di sindacato ispettivo in esame risale al maggio del 2008. Infatti, allora, il Ministero dello sviluppo economico convocò le prime riunioni invitando l'ex Eutelia a presentare il piano industriale. Nel gennaio 2009 l'azienda comunicò che il consiglio di amministrazione aveva deciso di focalizzare la propria attività sulle telecomunicazioni, uscendo dal settore delle tecnologie dell'informazione. Dopo diversi altri incontri susseguitisi con scadenza quindicinale, a giugno 2009 l'azienda Eutelia, pur convocata al tavolo di confronto del Ministero dello sviluppo economico, non si presentò a concludere la complessa trattativa le cui linee erano state, peraltro, condivise anche con il sindacato e, contestualmente, attuò la cessione del ramo d'azienda del settore informatico alla propria controllata Agile Srl, trasferendovi oltre 2.000 dipendenti. Dopo numerosi incontri svoltisi in varie sedi istituzionali in stretto raccordo con la Presidenza del Consiglio, preso atto delle dimissioni degli amministratori, il tribunale di Roma e il tribunale di Arezzo, verificati i presupposti, con due decreti del 14 luglio 2010, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 270 del 1999, hanno dichiarato rispettivamente

conseguente all'operazione di cessione del ramo d'azienda IT da Eutelia ad Agile e, peraltro, amplificata dalla sottoposizione di entrambe a una procedura concorsuale. In data 7 marzo sono stati approvati i programmi di cessione dei complessi aziendali facenti capo a entrambe le società.

che i programmi e le conseguenti procedure di vendita di Agile e Eutelia siano coordinate e finalizzate alla salvaguardia dell'unità operativa dei rispettivi complessi aziendali al fine di garantire, tramite lo sfruttamento di possibili sinergie tra i medesimi, la vendita combinata e/o integrata, per quanto possibile, delle attività e il maggior assorbimento occupazionale. Lo scorso 17 giugno il Ministro dello sviluppo economico, onorevole Paolo Romani, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1-*bis* (come introdotto dall'articolo 8, comma 3,

In data 12-13 luglio 2011 e, successivamente, il 1° settembre scorso i commissari straordinari hanno effettuato una pubblicazione congiunta del medesimo bando di vendita dei complessi aziendali redatto secondo i criteri dettati Il testo integrale del bando veniva reso, comunque, disponibile *on line* sui siti Internet delle due procedure. Il bando, nel prevedere la possibilità di offerta congiunta per più rami di azienda, riconosce un'adeguata premialità a quei piani industriali che assicurino un certo grado di complementarietà dei complessi aziendali Agile ed Eutelia, con preferenza per le soluzioni che garantiscano il minor impatto sociale da un punto di vista del mantenimento dei livelli occupazionali, una maggiore probabilità di salvaguardia degli *asset* industriali a elevata produttività e della maggior parte dei patrimoni aziendali. Preciso, infine, che in data 23 settembre scorso è scaduto il termine per la presentazione delle offerte di acquisto dei complessi aziendali Agile ed Eutelia e si è, pertanto, in attesa di conoscere l'esito della gara con la valutazione delle offerte pervenute. Quanto alla tutela dei lavoratori coinvolti, evidenzio che l'amministrazione straordinaria è affiancata da una specifica normativa in materia di ammortizzatori sociali, avvalendosi di una norma speciale (articolo 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236 del 1992). Con tale norma, per tutto il periodo di attività dei commissari, periodo che coincide con la durata del programma della procedura, viene garantita la Cassa integrazione guadagni straordinaria agli occupati. Solo a seguito della esecuzione del programma è possibile fare ricorso all'articolo 3 della legge n. 223 del 1991 recante norme in materia di cassa integrazione, mobilità e trattamenti di disoccupazione

altri 300 potrebbero andare in pensione. Ne rimangono 700 che hanno, in genere, dai 45 ai 55 anni. troppo giovani per andare in pensione e troppo vecchi, fra virgolette, per una diversa ricollocazione nel mercato. Da qualche parte, con l'aiuto delle Regioni e degli enti locali sono stati inseriti in progetti mirati di reinserimento, con formazioni specifiche e attività informatiche

E questo è il problema di questi lavoratori: un problema legato alla prima questione che le ponevo. Non basta avere una soluzione economica per la situazione di questa azienda che, peraltro, noi consideriamo tutt'altra e da non liquidare. una questione di piano industriale e di futuro. In secondo luogo, se noi distruggiamo un patrimonio che funziona, di fronte, purtroppo, a una crisi occupazionale che investe anche settori che devono essere riconvertiti, se distruggiamo un patrimonio altamente funzionante,

grave, e temo, viste le considerazioni che facevo sul "piccolo" Comune di Roma e su un paio di Ministeri, che vi sia anche una volontà politica

il settore della cantieristica, come noto, sta vivendo una fase di crisi internazionale molto pesante che ha determinato un crollo degli ordinativi a livello globale e una crescita della penetrazione commerciale dei cantieri asiatici, in particolare sulle navi da trasporto merci. La crisi ha avuto effetti molto negativi sui cantieri europei che hanno avviato una fase di profonda ristrutturazione con azioni di razionalizzazione della base produttiva - chiusura di cantieri - e consistenti riduzioni degli organici, valutabili in circa 40.000 occupati in meno, su un totale di circa 180.000. In questo contesto di forte difficoltà, il Governo italiano sta seguendo con grande attenzione l'evoluzione del settore, nella piena consapevolezza del ruolo fondamentale della cantieristica sull'industria nazionale, sia sotto il profilo del valore tecnologico del prodotto, sia sotto quello della rilevanza dell'indotto, in particolare in alcune aree del Paese. Per affrontare tempestivamente gli effetti della crisi internazionale, il Governo italiano sta operando sia con iniziative autonome, sia in raccordo con le iniziative della Commissione europea, a difesa del settore. A livello nazionale è stato istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, fin dal 2008, un tavolo di confronto con tutte le parti interessate che ha portato alla sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa del dicembre 2009. Rispetto agli impegni assunti dal Governo nel protocollo, nonostante le note difficoltà finanziarie, in questi due anni sono stati fatti significavi passi in avanti. L'accordo tra Cassa depositi e prestiti e SACE ha consentito a Fincantieri di acquisire importanti commesse nel segmento *cruise*. La Fincantieri ha perfezionato l'acquisizione della seconda nave Carnival, delle quattro previste dall'accordo quadro, per un valore di 800 milioni di Euro. Coerentemente con quanto previsto dal protocollo, è stata assegnata dal Governo la commessa per due pattugliatori per le Capitanerie di porto, per la quali è stata ultimata la progettazione ed è iniziato il «taglio della lamiera», consentendo un carico di lavoro per il cantiere per circa due anni, con una media di 250 occupati. Per quel che riguarda, invece, l'avvio del progetto relativo alle navi multiruolo e logistiche per la protezione civile e per la Marina militare, il Governo ha confermato l'impegno a stanziare le risorse necessarie per la progettazione Sul fronte del sostegno alla ricerca, che rappresenta la principale leva per garantire la competitività del settore, il Ministero dello sviluppo economico ha finanziato, nell'ambito del progetto «Industria 2015», due progetti, presentati da Fincantieri in collaborazione con piccole e medie imprese e centri di ricerca, per la realizzazione di sistemi e impianti di bordo innovativi e

l'iniziativa "Ritmare" con un finanziamento deliberato dal CIPE di 450 milioni di euro. Il progetto prevede, tra l'altro, la realizzazione di navi oceanografiche e lo sviluppo di altre tecnologie marittime. È infine già operativa la piattaforma tecnologica nazionale marittima, che coinvolge i Ministeri interessati, i cantieri, gli armatori e i centri di ricerca del A livello europeo il Governo italiano sta sostenendo l'azione intrapresa dal vice presidente Antonio Tajani mirata a dare nuovo impulso alla strategia europea a sostegno della riqualificazione del settore. In particolare, la Commissione si sta muovendo lungo tre direttrici: rilancio del ruolo della BEI nei finanziamenti alla cantieristica, confermando il vincolo "UE *built*" e introducendo la possibilità di estendere il finanziamento anche ad armatori operanti fuori dall'Unione; l'estensione al 2020 del programma "Leadership 2015", che prevede la possibilità di concedere aiuti al settore per attività di ricerca e sviluppo e per la costituzione di un fondo europeo di garanzia per gli investimenti pre-*delivery*; definizione di un quadro di riferimento europeo per la rottamazione dei traghetti, finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale delle attività marittime. In esito al confronto che si sta sviluppando in Europa, il Governo italiano adotterà misure coerenti con gli indirizzi che saranno assunti in sede comunitaria. In relazione alla bozza di piano industriale presentata dalla Fincantieri ai sindacati nell'incontro del 23 maggio scorso, che annunciava la chiusura di due cantieri e ampie riduzioni occupazionali, il Governo, dando immediata risposta alla richiesta delle organizzazioni sindacali, ha convocato il tavolo della cantieristica il 3 giugno. In quell'occasione il ministro Paolo Romani ha preso atto della decisione dell'azienda di ritirare la bozza di piano industriale e della necessità di affrontare le criticità presenti in alcune aree. Conseguentemente, il Ministro ha invitato l'azienda a ricercare nuove soluzioni industriali e nuovi modelli organizzativi, prendendo anche in esame la possibilità di aggredire nuovi mercati e di sviluppare nuovi prodotti. Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre assunto l'impegno di istituire immediatamente tavoli di confronto con le Regioni interessate ai più importanti interventi infrastrutturali che riguardano anche i cantieri di Castellammare di Stabia in Campania. Per quel che riguarda la Campania, il MISE ha avviato con la Regione, la Provincia di Napoli, il Comune di Castellammare di Stabia e l'autorità portuale, la discussione propedeutica alla sottoscrizione di un protocollo di intesa per il rilancio produttivo e occupazionale del cantiere e dell'indotto. La firma dello stesso è prevista entro la prima metà del mese di ottobre. In ogni caso, questo intervento, oneroso per il Paese, dovrà garantire l'occupazione e la difesa delle professionalità presenti nelle diverse aree. Infine, per affrontare la questione degli ammortizzatori sociali, il Governo si è impegnato ad attivare presso il Ministero del lavoro un tavolo per la definizione delle necessarie proroghe della cassa integrazione cantiere per cantiere. In conclusione, il Governo è pienamente consapevole della necessità di avviare un processo di rafforzamento e di riorientamento della cantieristica italiana al fine di garantire una stabile competitività sui mercati internazionali. Tale processo, necessario per far fronte alle trasformazioni imposte dalla crisi globale del settore, deve però essere inserito in un quadro di politiche europee e nazionali condivise con le organizzazioni sindacali e con le istituzioni locali.

Il Governo ha dato quattro risposte - la sua è la quarta - molto simili tra loro,

lei ha fatto riferimento alla giornata del 3 giugno, durante la quale, grazie al grande impegno dei lavoratori e del sindacato, quel piano scellerato presentato dall'azienda, che prevedeva la chiusura dello stabilimento di Castellammare, è stato ritirato. In quell'occasione, il Ministro dello sviluppo economico prese impegni precisi: assicurò che sarebbe stato chiesto all'azienda di redigere un nuovo piano industriale; che si sarebbero istituiti due tavoli, uno per la regione Liguria e l'altro per la regione Campania; che ci sarebbe stato il prosieguo della cassa integrazione. il tavolo per la Campania non è mai stato istituito: non ha mai lavorato ad un progetto industriale.

per l'ammodernamento del cantiere di Castellammare, procedere al finanziamento del bacino di costruzione: anche di questo non si è più manca un'ipotesi definitiva in tal senso. Voglio ricordare che la questione riguarda oltre 2000 lavoratori, tra i dipendenti e l'indotto.

l'azienda, davanti alle istituzioni locali e ai rappresentanti del Governo, ha presentato a Napoli il progetto «Plasmare» per la realizzazione di impianti navalizzati per il trattamento dei rifiuti solidi urbani. Si tratta di piattaforme, che secondo il progetto dovrebbero contenere i rifiuti, una sorta di CDR galleggianti.

Tuttavia, non si conosce la tempistica. Lo stesso direttore, dottor Bono, amministratore delegato di Fincantieri, ha sottolineato, nella presentazione di questo progetto, che c'è un problema di adeguamento tecnologico: un progetto quindi non immediatamente cantierabile. Non si fa il bacino di costruzione, non si fa l'adeguamento tecnologico per cantierare questo possibile progetto, non esiste un nuovo piano industriale Fincantieri a seguito del ritiro dell'altro piano; non è stato convocato un altro tavolo che veda intorno tutti gli interlocutori e protagonisti di questa vicenda.

si arrivi alla definizione di commesse da dare a Fincantieri-Castellamare di Stabia, ma anche di questo si perde traccia. questione, come tutta la questione della grave crisi industriale che attraversa la regione Campania, debba essere affrontata con serietà, concretezza

parte da Fincantieri, ma anche da altre questioni drammatiche che qui sono state portate in discussione, da Irisbus ad Ansaldo Breda, ed altre.

questo Ministero può e vuole contribuire alla piena tutela della maternità implementando programmi di prevenzione nell'area della salute della donna e della tutela della maternità, per attuare i quali un importante strumento è costituito dal consultorio familiare. finalità comune per il Ministero della salute e per le Regioni è la piena sintonia dì intenti volti ad aiutare la donna a superare le cause che potrebbero indurla all'interruzione di gravidanza (intervento peraltro previsto dalla legge n. tramite interventi dì natura sociale e sociosanitaria integrata o, nel caso in cui questo non fosse possibile, seguendo adeguatamente la donna nell'intero percorso, sia da un punto di vista medico che psicologico. Ogni Regione provvede autonomamente, attraverso i servizi consultoriali, alla gestione di progetti che spesso vedono coinvolte associazioni di volontariato. Il Ministero della salute ha supportato e finanziato progetti che mirano a ridurre i tassi del ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza tra le donne, italiane e straniere, attraverso la promozione di una maggiore consapevolezza della loro salute, una maggiore conoscenza dei metodi utili ad una procreazione cosciente e responsabile, la formazione di operatori sociosanitari, la diffusione della conoscenza delle norme a sostegno della maternità e contro l'abbandono dei neonati. Le istituzioni centrali e regionali hanno come compito il governo del sistema, per la riduzione progressiva dell'incidenza del fenomeno, per l'abbattimento dell'aborto clandestino, per la promozione della procreazione consapevole, al fine di evitare che l'aborto divenga un mezzo per il controllo delle nascite. Segnalo, in particolare, che lo schema di piano sanitario nazionale 2011-2013, di cui è prossima l'approvazione finale, pone tra le priorità del Servizio sanitario nazionale la tutela della donna durante tutto il percorso nascita (dalla fase preconcezionale al puerperio) e quella del nascituro. In tale ambito, è possibile il miglioramento del grado di integrazione in rete dei servizi di 1° livello (consultori familiari, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta), 2° livello (poliambulatori distrettuali e ospedalieri), 3° livello (centri nascita a diverso grado di complessità), nonché la razionalizzazione dei punti nascita. Lo stesso piano individua, tra le criticità da affrontare, la carenza di informazioni e di conoscenze fra le donne, e, in particolare, fra le madri con bassa istruzione o straniere. Proprio a queste ultime è stato dedicato un progetto, finanziato nel 2010 dal Ministero della salute attraverso il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, finalizzato a prevenire il ricorso all'IVG e a migliorare l'accesso alle informazioni sui servizi sociosanitari dedicati all'area materno-infantile, come i consultori, e sulle norme a sostegno della maternità e contro l'abbandono dei neonati. Le principali aree di intervento sono tre: la formazione degli operatori sociosanitari ad un approccio interculturale delle prestazioni; la definizione e la sperimentazione di percorsi organizzativi che favoriscano l'accessibilità e l'utilizzo dei servizi da parte delle donne immigrate; la promozione di una diffusa informazione per la popolazione immigrata finalizzata alla tutela della salute materno-infantile e alla prevenzione dell'aborto. Il progetto, tutt'ora in corso in otto Regioni, coinvolge le aziende sanitarie locali e le società scientifiche ma soprattutto i mediatori culturali e le associazioni di immigrati più rappresentative del territorio che contribuiscono, ciascuna attraverso la propria rete informale di contatti, a una più capillare distribuzione del materiale informativo realizzato. Voglio ricordare che da molti anni ormai il tasso di abortività nel nostro Paese continua a scendere e che effettivamente il tasso di abortività fra le immigrate è ormai il vero dato preoccupante fra quelli che raccogliamo ogni anno per la relazione al Parlamento. Segnalo, altresì, che il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, in stretta collaborazione con l'associazione di promozione sociale Movimento per la vita italiano, la comunità Papa Giovanni XXIII e l'associazione Ai.Bi.-Amici dei bambini, ha ideato un progetto sperimentale dal titolo: «Adozione: un'alternativa all'aborto». In particolare, il Dipartimento e il consorzio Preferire La Vita, costituito tra le tre citate associazioni, si sono impegnati, per i prossimi due anni, nella realizzazione di tale iniziativa, volta a promuovere la tutela della maternità e della vita nascente anche attraverso la pratica del parto in anonimato, ove non vi siano altre alternative. Scopo dell'iniziativa è promuovere fattivamente e culturalmente, come valore positivo in alternativa all'aborto, la nascita del figlio non atteso, offrendogli l'opportunità di essere accolto e amato dalla stessa mamma, opportunamente aiutata da un'altra famiglia idonea ad accoglierlo e amarlo come un figlio proprio. Gli interventi promossi dal citato consorzio si realizzeranno attraverso la capillare rete di oltre 500 sedi territoriali e locali diffuse sul territorio nazionale. Alcuni di tali interventi attengono proprio all'«area ascolto all'«area ascolto e informazione», nell'ambito della quale sono inserite tutte le attività volte a informare le gestanti sulle possibilità che il consorzio offre, nonché a raccogliere le domande di aiuto e le attività di orientamento verso il percorso maggiormente rispondente al bisogno rilevato. della salute è assolutamente concorde sulla necessità che tutte le istituzioni pubbliche, nell'ambito delle proprie specifiche competenze, pongano in essere gli interventi più idonei affinché la legge n. 194 del 1978 sia attuata in tutte le sue parti, in particolare nella prima parte che riguarda la prevenzione e la tutela della maternità. A tal fine, le attività di informazione circa le strutture pubbliche e le associazioni del privato sociale esistenti sul territorio volte ad aiutare e ad accogliere le donne in gravidanza, e in particolare sui consultori e sulle loro funzioni, assumono particolare importanza.

Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, è di tutta evidenza che questa interrogazione, presentata il 15 settembre 2010, era una una provocazione: non avevo citato nemmeno chi era l'operatore che aveva dato quel consiglio, perché si trattava esattamente di fare in modo che, attraverso tutte le strutture possibili e immaginabili, con i compiti propri delle istituzioni e con l'apporto del volontariato, si divulgasse la notizia che

tutto sommato mettendo sulle spalle della donna ed eventualmente della sua famiglia un'attività di welfare, mi interessava che si verificasse

quali sono i risultati che si ottengono esattamente con ciò che lei ci ha illustrato alla fine del suo intervento: il consorzio, come agisce, su quante persone lavora, che risultati si ottengono. In questa maniera si difende anche la legge n. 194, perché effettivamente chi le parla non l'ha votata, ma quando una legge dello Stato va attuata in tutte le sue parti; gli strumenti citati possono essere certamente funzionali e coerenti con la parte che deve prevenire il ricorso all'aborto aiutando la mamma e le famiglie italiane in genere. Quindi, sarei

evidenzio come le suddette finalità promozionali siano riferite prevalentemente ai prodotti commercializzati dal marchio menzionato e non siano, di fatto, riconducibili alla promozione di nessuna figura professionale, anche se bene avrebbe fatto l'articolo in questione a indicare la professione sanitaria del podologo

alla luce delle premesse di cui sopra, non integrano un'ipotesi di pubblicità sanitaria ingannevole, unica fattispecie nella quale è consentito intervenire ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 2006, n. 248.

così parziali e di nicchia, perché si tratta di una di quelle professioni sanitarie non mediche che vanno tutelate, nel senso di garantire ai cittadini che sia effettivamente una professione sanitaria e non estetica, come potrebbe essere quella del pedicure. Il piede è troppo importante, in tutte le fasi della vita, ma, se penso ai bambini e agli anziani, un'accurata assistenza preventiva e curativa significa, per gli anziani, qualche volta evitare l'allettamento

certamente il Ministero, attraverso i NAS, fa un'opera molto meritevole (e lo ribadisco in questa sede, per esprimere anche la nostra gratitudine), mi corre l'obbligo di fare in modo, siccome il Parlamento è impegnato, sia alla Camera che al Senato, su figure, professioni, albi, ordini, cioè su misure e norme da migliorare, da integrare o da innovare, che questa professione sia tenuta in debita considerazione, proprio per la sua utilità rispetto al benessere delle persone.

al medico chirurgo specializzato in odontoiatria come potrebbe stare il podoiatra alla figura dell'ortopedico. Sarebbe un modo per alleggerire le facoltà, fare in modo che le specializzazioni diventino più affinate e che ci siano professioni equivalenti a quelle degli altri Paesi. Infatti, onorevole Sottosegretario, lei sa che le nostre frontiere, giustamente, sono penetrabili quando ci sono professioni sanitarie di altri Paesi - penso alla Spagna che ha il podologo e il podoiatra - che potrebbero oggettivamente favorire una migrazione di professionisti che vengono da un altro Paese quando, invece, anche in Italia potremmo offrire ai giovani, come professione, e ai cittadini, come utenti di un sistema sanitario che integra prevenzione, cura e riabilitazione, figure meno medicalizzate e meno costose che però creano vantaggi oggettivi al sistema sanitario e alla tutela della salute del singolo.

La rete è composta da 19 Banche operative, collocate in 13 Regioni italiane. Alle Banche sono collegati circa 300 punti nascita sul territorio nazionale, dove è possibile effettuare la donazione di sangue cordonale. L'inventario nazionale è, ad oggi, costituito da un numero complessivo di 32.192 unità cordonali, donate in modo volontario, anonimo e gratuito per l'impiego terapeutico nel trapianto allogenico di midollo osseo da donatore non consanguineo, quale fonte alternativa di cellule staminali emopoietiche per pazienti, adulti e pediatrici, che non trovano donatori adulti compatibili nell'ambito familiare e dei registri nazionale ed internazionali dei donatori volontari di midollo osseo. La Banca di Sciacca, in conseguenza delle vicende che hanno riguardato la precedente gestione, ha sospeso le attività nel 2006 e le ha riprese nel 2008, dopo essere stata sottoposta a visita di verifica da parte delle autorità sanitarie regionali e del Centro nazionale sangue, di concerto con il Centro nazionale trapianti, su mandato del Ministero della salute. Dalla visita di verifica sono emerse la necessità di apportare al sistema organizzativo della Banca consistenti azioni correttive, al fine di renderlo adeguato agli *standard* vigenti e di consentire alla stessa Banca di partecipare attivamente alla composizione dell'inventario nazionale delle unità di sangue cordonale; la necessità di operare una riqualificazione dell'inventario preesistente, composto dalle unità cordonali raccolte prima del 2006, in quanto patrimonio biologico di valenza nazionale. La Banca di Sciacca, grazie a un finanziamento a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione di progetti obiettivo di Piano sanitario nazionale per l'anno 2010 (accordo Stato-Regioni dell'8 luglio 2010), ha potuto avviare nel 2011 il percorso della riqualificazione di taluni lotti di unità cordonali già criopreservate. In particolare, le risorse messe a disposizione fino ad oggi (tenuto conto anche delle risorse vincolate in tema di «Interventi a favore delle biobanche di materiale umano» di cui all'accordo Stato-Regioni del 25 marzo 2009) dalla Regione Sicilia sono state impiegate per: realizzare il piano delle azioni correttive richiesto dagli organismi regionali e nazionali competenti; riprendere le attività di raccolta e crioconservazione delle unità cordonali con modalità totalmente aderenti agli standard vigenti; ottenere l'autorizzazione da parte delle autorità nazionali competenti ad esporre le unità cordonali crioconservate presso lo Sportello unico nazionale avviare uno studio di fattibilità per la riqualificazione delle unità cordonali bancate negli anni precedenti. Dalla ripresa delle attività, avvenuta nell'aprile 2008, al 31 dicembre 2010, la Banca ha raccolto 3.333 unità cordonali da donatrici volontarie e 282 unità cordonali dedicate. delle unità cordonali donate a scopo solidaristico sono state bancate perché perfettamente rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza necessari per l'impiego trapiantologico. L'indice di bancaggio (rapporto tra unità raccolte e unità effettivamente bancate) della Banca di Sciacca del 24 per cento è del tutto sovrapponibile all'indice medio nazionale, a dimostrazione che la Banca sta operando in totale conformità ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici, definiti con apposito accordo Stato-Regioni del 29 ottobre 2009 e adottati dalla rete italiana delle banche di sangue cordonale. La Banca di Sciacca sta inoltre applicando, per il bancaggio delle nuove unità cordonali, criteri qualitativi e quantitativi del tutto conformi a quelli stabiliti dal *network* italiano e dagli *standard* internazionali applicabili. La Banca di sangue cordonale di Sciacca non ha ancora ripreso le attività di rilascio delle unità cordonali per trapianto allogenico non familiare ai centri trapianto italiani ed esteri; tali attività sono invece già riprese per le unità cordonali conservate a scopo dedicato. D'altra parte, il rilascio di unità cordonali nell'ambito dei circuiti nazionali e internazionali di trapianto allogenico di cellule staminali emopoietiche è subordinato alla presenza di requisiti organizzativi certificati, che la Banca sta progressivamente conseguendo attraverso il piano delle azioni correttive. In relazione alle attività necessarie per il recupero delle unità cordonali raccolte prima della chiusura della Banca (circa 20.000 unità), il direttore del Centro nazionale sangue ha ricevuto, con decreto assessoriale 2084 del 12 agosto 2010, il mandato di realizzare, all'interno del complessivo progetto di riqualificazione della Banca stessa, un piano di recupero sostenibile delle unità crioconservate prima del 2006, sotto la guida di una consulenza specialistica proposta dal CNS e scelta in conformità alle indicazioni del decreto ministeriale 18 novembre 2009 («Istituzione di una rete nazionale di banche di sangue del cordone ombelicale»), che individua la Banca di sangue cordonale della Regione Lombardia quale ente di riferimento tecnico-operativo della rete nazionale. Il piano di riqualificazione prevede una sequenza di azioni volte a verificare, progressivamente e secondo criteri di costo/efficacia, la qualità, la sicurezza e la tracciabilità delle unità cordonali, che costituiscono l'inventario pregresso, al fine di recuperare e rendere patrimonio di tutto il *network* italiano solo quelle unità che rispondano completamente ai requisiti cogenti e ai parametri qualitativi e di sicurezza indispensabili per entrare nell'inventario nazionale e mondiale. La prefettura-ufficio territoriale del Governo di Agrigento ha segnalato che in sede regionale risultano essere stati adottati interventi a supporto delle attività proprie della Banca del sangue cordonale di Sciacca, al fine di assicurare la piena operatività della biobanca, l'esposizione delle unità cordonali prelevate negli anni più recenti e la fruibilità dei prodotti raccolti nel periodo antecedente il 2006, laddove risulteranno conformi ai cogenti requisiti richiesti dalla normativa di settore. È auspicio - e interesse - del Ministero della salute che in futuro possa consolidarsi la collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali competenti, e in primo luogo la Regione Sicilia, al fine di migliorare ulteriormente il livello di qualità della Banca cordonale di Sciacca,

Presidente, signora Sottosegretario, mi ritengo parzialmente soddisfatto dalla lettura della risposta che gli uffici le hanno preparato, perché condivido l'importanza strategica della funzione della Banca ombelicale, l'importanza strategica della messa in rete delle banche la capacità di offrire un servizio avanzato in un settore di nicchia ma strategico e importante, in grado di offrire realmente al nostro Paese degli standard elevati. Nello stesso tempo, signora Sottosegretario, rimprovero un ritardo nella risposta. Questa interrogazione è stata fatta il 3 agosto del 2010, rimbalzo questo «rimprovero» all'attenta riflessione della nostra Presidenza, per evitare che le sollecitazioni e le osservazioni che avanziamo siano poi sfasate rispetto alle risposte che qui ci vengono offerte. Prendo inoltre atto che ci sono state un'attenzione nell'ultimo periodo e una cura un po' diversa rispetto al passato. Quando ho fatto l'interrogazione, il rischio era che si perdesse

in grado di svolgere una funzione molto importante per rendere disponibile almeno una parte del capitale biologico criopreservato a scopo di trapianto, a favore dei pazienti eleggibili.

l'assessore Russo ha avuto il coraggio di applicare la legge. In poche Regioni d'Italia si guarda agli *standard* e alla capacità di rispettare gli obiettivi e il *budget*. Oggi il vecchio dirigente generale non c'è più: c'è un nuovo commissario. La prego pertanto, onorevole Sottosegretario, di prestare sempre cura e attenzione per verificare se si provvederà ad alimentare la giusta sinergia e di non fare, anche nelle risposte, allusioni pregiudizievoli nei confronti di chi oggi in Sicilia, nella gestione della sanità, sta ottenendo delle *performance* senza precedenti, sia in termini di contenimento di costo (la regione Sicilia non fa parte più della

ha dichiarato di essere accreditato con il Servizio sanitario nazionale e, quindi, di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal regolamento regionale n. 14 del 30 giugno 2009, avente ad oggetto 3, comma 1, lettera a), punto 1) della L.R. 28 maggio 2004, n. 8. Determinazione degli ambiti territoriali e fabbisogno prestazioni PET per il rilascio della verifica di compatibilità e dell'accreditamento istituzionale alle strutture sanitarie e socio-sanitarie». A tale proposito, l'assessore regionale alle politiche della salute ha precisato che: l'accreditamento istituzionale attiene alla fase conclusiva del procedimento avviato con il rilascio, da parte del competente servizio, della verifica di compatibilità, a seguito di istanza del Comune territorialmente competente; il regolamento regionale n. 14 del 30 giugno 2009 individua, all'articolo 4, lettera b), il fabbisogno regionale di una PET da installare presso strutture sanitarie private, per ciascun ambito territoriale pari o superiore a 750.000 abitanti, purché in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di medicina nucleare, rilasciata ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2004. Nel merito del quesito, il giorno 18 marzo 2011 si è riunita, presso l'assessorato alle politiche della salute della Regione Puglia, la Conferenza dei servizi per trattare l'argomento riguardante le problematiche di competenza del Sistema sanitario della Regione Puglia e le prestazioni PET/TC a cui hanno preso parte i rappresentanti del Centro di medicina nucleare Calabrese, In tale sede i partecipanti hanno convenuto di ripercorrere l'*iter* amministrativo finalizzato alla verifica, da parte della stessa Regione, dei requisiti per la erogazione delle prestazioni di medicina nucleare/Pet Tac ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Con il provvedimento n. 83 del 2011 l'assessorato alle politiche della salute ha autorizzato l'esercizio dell'attività di medicina nucleare con erogazione di PET/TC al «Centro di medicina nucleare Calabrese». Proprio in data 26 settembre 2011 è stato firmato il provvedimento regionale di accreditamento,

non sono Vendola e quindi parlo semplicemente di schizofrenia, rispetto a un modo di fare che veramente non si comprende. Anche perché nella sua risposta, signora Sottosegretario, lei arriva alla conclusione dopo due anni, perché la pratica è iniziata niente meno che nel gennaio del 2008, e finalmente, trascorsi due anni, la Regione Puglia

è stato eletto. Ricordo che nel 2009 la Regione Puglia ha dovuto affrontare costi per oltre 2 milioni di euro per remunerare le prestazioni di PET/TAC effettuate dai malati oncologici salentini - solo da questi - nelle diverse strutture sparse su tutto il territorio nazionale. Ricordo anche che nel 2011 ha speso ben 2.056.905,31 per essere precisi - sempre per lo stesso motivo, perché questi ammalati (e naturalmente le famiglie, con tutto ciò che comporta il cosiddetto viaggio della speranza verso altre Regioni) si sono dovuti recare: 10 in Piemonte, 279 in Lombardia, 31 in Veneto, 1 in Liguria, 149 in Emilia-Romagna, 11 in Toscana, 2 in Umbria, 106 nel Lazio, 2 in Abruzzo, 267 in Campania, 942 in altre province pugliesi e 147 in Basilicata. Inutile ricordare che tutte le prestazioni debbono essere remunerate a costo pieno dalla ASL di Lecce alle strutture eroganti. Quindi, non capisco quale convenienza vi sia stata per per il presidente Vendola e per il suo assessore alla sanità nello spendere oltre 2 milioni di euro per il 2009 e altrettanti per il 2010.

situazione - il giudice di pace, su richiesta di cinque malati oncologici e su pressione del Codacons ha convocato il presidente Vendola perché testimoni sulle ragioni per le quali l'amministrazione regionale costringe i malati oncologici salentini ad affrontare i cosiddetti viaggi della speranza. Mi permetto di ricordare ancora, in questa sede, che faccio parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sull'efficacia e l'efficienza - si fa per dire - del Servizio sanitario nazionale nazionale e che in questa Commissione il primo *focus* è stato acceso proprio sulla sanità della regione Puglia, della quale, peraltro, si parla tantissimo,

per andare a fondo, e non per una curiosità del sapere, ma semplicemente perché è un dovere, da parte di un parlamentare, cercare di comprendere il motivo per il quale, nella propria regione, si spendono inutilmente tanti danari e si è poi costretti ad aumentare le tasse

del Senato per dire che, purtroppo, è molto deludente la risposta che fino ad oggi, dopo tre anni dall'insediamento della Commissione, è stata data in merito a questa tematica. Una tematica regolarmente messa da parte, e che ha visto soltanto una relazione da parte del relatore. Ho sollecitato una risposta più volte, attraverso una serie di documenti che ho fornito, documenti ufficiali, di stampa, senza nessun aspetto scandalistico - eppure ce ne sarebbe forse motivo